presentate dai lavoratori ai fini della formazione di una graduatoria per accedere al contributo *una tantum*, previsto dalla legge regionale 18 maggio 2007, n. 10, recante «Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto», diretto ad assicurare, per limitati

A tale proposito, come già evidenziato nella risoluzione n. 193/E del 2008, l'Agenzia delle entrate ricorda che il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sulla possibilità di esenzione dal bollo delle domande preordinate all'ottenimento di provvidenze e contributi, in relazione a quanto disposto dal predetto articolo 8, comma 3, ha precisato che «Sussistono motivi di perplessità per poter effettivamente superare la prassi consolidata seguita dall'amministrazione finanziaria in base alla quale [...] il beneficio dell'esenzione in parola è stato applicato esclusivamente alle istanze relative alle richieste di sussidi delle persone non abbienti Non sembra di secondario rilievo la circostanza che la prevista esenzione relativa alle domande per "sussidi" venga associata, nella stessa norma, ad altra ipotesi concernente le domande "per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti" [...]. Oltretutto non va dimenticato che il limitato ammontare dell'imposta di bollo giustificherebbe l'esenzione soltanto se a favore di persone effettivamente indigenti, tenuto anche conto del carattere indiscriminato ed uniforme di tale forma di imposizione tributaria, destinata per sua natura a colpire nello stesso modo la generalità dei soggetti che versino in determinate situazioni, senza di norma operare distinzioni in relazione a condizioni soggettive anche precarie dei soggetti stessi». Questo è il parere del Consiglio di Stato, sezione III, del 13 maggio 1997, n. 656. In definitiva, seppur la finalità del contributo previsto dalla legge regionale veneta n. 10 del 2007 è di garantire ai cittadini prospettive di sicurezza economica al termine dell'attività lavorativa ed alleviare loro un possibile disagio sociale, non sembra che lo stesso sia assimilabile alle ipotesi disciplinate dall'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al decreto del Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'Agenzia delle entrate ritiene che le norme in vigore disciplinanti la materia in trattazione non consentano di escludere dall'applicazione dell'imposta di bollo le domande presentate al fine di ottenere i benefici di cui alla legge regionale veneta n. 10 del 2007.

conclusione cui arriva il Ministero, anzitutto perché stiamo parlando di una specifica attività promozionale per fare in modo che coloro che hanno particolari tipologie lavorative

credo sia utile ricordare che la previdenza complementare è stata istituita con un meccanismo di grandi agevolazioni fiscali proprio per renderla per incentivarla. Infatti, questo istituto - che ancora incontra grandi resistenze nel nostro Paese, soprattutto da parte delle giovani generazioni

possibilità per costruire, in prospettiva, alla fine della vita lavorativa, un trattamento previdenziale che non li faccia dipendere dall'assistenza pubblica. Lei sa, signor Sottosegretario, che quando si arriva alla fine della vita lavorativa e la pensione

la novità e la modernità della vostra concezione dello Stato sociale, basata sull'iniziativa individuale e sull'intervento pubblico. Se sono le norme che impediscono di avere

Gli onorevoli interroganti, nel far presente che sarebbero state notificate ai cittadini circa 1,6 milioni di cartelle esattoriali sbagliate, chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare per risolvere il fenomeno delle cosiddette cartelle pazze e per tutelare i contribuenti. A tale riguardo, l'Agenzia delle entrate ha osservato, in via preliminare, che la riforma del sistema della riscossione nazionale dei tributi, con il conseguente passaggio del servizio stesso ad Equitalia spa, ha prodotto effetti positivi sia in termini di incremento dei volumi della riscossione e, quindi, di contrasto all'evasione fiscale, sia in termini di miglioramento del servizio offerto ai cittadini e alle imprese, rispetto a quello offerto dagli ex concessionari della riscossione, ovvero le banche. Per quanto concerne, in particolare, le difficoltà che i contribuenti avrebbero riscontrato nel contattare direttamente la società Equitalia, i competenti uffici di Equitalia, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, hanno fatto presente che sono molteplici le iniziative intraprese e quelle in corso di realizzazione per migliorare i servizi ai contribuenti. Si tratta, in particolare, della razionalizzazione della rete territoriale degli sportelli (circa 380, oltre a 15 sportelli dedicati e ai 26 presenti all'interno degli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS), della stipulazione di convenzioni con ordini professionali, nonché della diffusione capillare della guida pratica per il cittadino-contribuente, contenente informazioni e indicazioni utili ai cittadini che ricevono una cartella di pagamento. Inoltre, dal 4 novembre 2008 è stata attivata, contestualmente alla pubblicazione dei nuovi siti del gruppo Equitalia, la casella di posta elettronica che consente di chiedere e ricevere direttamente informazioni. Infine, è in corso di studio la realizzazione di un numero telefonico unico, che consenta il contatto diretto telefonico con l'Agente della riscossione in modo da rispondere alle legittime aspettative dei contribuenti. Relativamente alla notizia diffusa da organi di stampa e media, secondo cui sarebbero state emesse in in sei mesi circa 1.600.000 cartelle pazze, la società Equitalia ritiene di dover smentire tale dato in quanto, come risulta dalle informazioni in proprio possesso ottenute dal monitoraggio delle società partecipate del gruppo, non esiste un fenomeno così vasto Infatti, da tale monitoraggio, emergerebbe una percentuale di contestazioni sull'operato di Equitalia pari all'1,24 per cento di ricorsi, a fronte di oltre 17 milioni di atti emessi, con un indice di errore inferiore allo 0,5 per cento, come riscontrato dai dati forniti da alcuni agenti della riscossione operanti in significative aree territoriali. Comunque, l'Agenzia delle entrate ed Equitalia stanno procedendo celermente possibile in questa opera di modernizzazione del sistema e di rapporto diretto con il contribuente. Obiettivo di questo Governo è velocizzare e migliorare

far rizzare i capelli. Comunque, anche la modalità con cui Equitalia sta migliorando i tempi di risposta e il servizio non ci trova pienamente d'accordo.

ispettivo in esame gli interroganti hanno chiesto di conoscere quali iniziative si intenda assumere riguardo alla proprietà del nuovo argine di conterminazione lagunare, dello specchio acqueo e della viabilità relativa, siti in Quarto d'Altino (in provincia di Venezia), che risulterebbe di proprietà della società Vivaldi srl. Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha rappresentato che, ad oggi, la società Vivaldi srl non ha ancora ceduto la proprietà di cui trattasi, in quanto pende, innanzi al tribunale ordinario di Venezia, un procedimento civile promosso dalla predetta società nei confronti del Magistrato alle acque di Venezia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Agenzia del demanio - con estensione successiva del contraddittorio anche nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - per l'accertamento della proprietà privata dei luoghi predetti in capo alla società. E finché il procedimento pendente non sarà chiuso, non sarà possibile chiarire quanto

anche questa risposta purtroppo non ci soddisfa pienamente. Sarà pur vero che c'è un procedimento civile in corso, ma questo trasferimento di proprietà tra privati di un bene demaniale - anche qui poi bisognerebbe capire come abbia fatto un notaio a sottoscrivere un simile atto, ma questa è un'ulteriore questione

comporta un danno ambientale tuttora in corso. Almeno su questi aspetti bisognerebbe procedere con tempi più rapidi di quelli della magistratura.

non è per la percentuale di votazione, che riteniamo essere un modo ridicolo per valutare il lavoro dei parlamentari, ma per il concetto stesso di appartenenza all'Assemblea non riteniamo né giusto né opportuno che,